Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Piemonte, a seguito della morte del senatore Ugo Martinat, ha riscontrato che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Tomaso Zanoletti. Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Tomaso Zanoletti. *(Applausi dal

reclami. La figura del senatore Martinat sarà ricordata nel corso della seduta pomeridiana di domani, alle ore 17. comunico, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti è convocata, per procedere alla sua costituzione domani, mercoledì 1° aprile,

*(PD)*. Signora Presidente, ho chiesto la parola perché, come lei sa, nella giornata di ieri è avvenuta una tragedia immensa, della quale non siamo ancora in grado di misurare le dimensioni:

parola. La informo comunque che la Presidenza è già in contatto con il Governo perché l'Esecutivo decida al più presto in quale formula e in quale sede intende riferire al Parlamento, in

il contenuto del disegno di legge d'iniziativa del senatore Centaro. Il risultato dell'esame in Commissione, nel corso del quale sono state svolte anche alcune audizioni informali di associazioni che si occupano di usura,

A distanza di oltre dieci anni, crediamo sia giunto il momento di risolvere alcune criticità che queste leggi hanno manifestato nell'applicazione pratica. Il Capo II, invece, è particolarmente innovativo perché introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento,

per l'erogazione dei mutui concessi alle vittime dell'usura dall'apposito Fondo di solidarietà e, dall'altro, modificando la composizione della Commissione preposta alla gestione di tale Fondo. L'articolo 2 interviene, poi, sulla legge 23 febbraio 1999, n. 44, precisando il concetto di evento lesivo, presupposto essenziale per l'elargizione a favore dei soggetti vittime di attività estorsive, consentendo la cumulabilità con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche, modificando i criteri per la individuazione dei soggetti rappresentativi di associazioni od organizzazioni facenti parte del comitato di solidarietà e, infine, modificando le norme in materia di sospensione di termini. Con l'articolo 3 si è intervenuti sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007, in materia di confidi, ribadendo il mantenimento dei vincoli di destinazione per i soggetti beneficiari del contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Con gli articoli 4 e 5 sono state apportate alcune significative modifiche al codice penale. In particolare, con l'articolo 4, si è integrato l'articolo 629 del codice penale in materia di estorsione, prevedendo quale aggravante di pena anche l'ipotesi in cui il fatto estorsivo sia commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari, mentre, con il successivo articolo 5, si è modificato l'articolo 644 del codice l'affidamento al giudice della decisione di restituire o meno i titoli, i beni e le utilità

è l'articolo 6, che ha modificato il comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e con il quale è stata esclusa l'applicabilità della pena su richiesta delle parti anche per i reati di estorsione ed usura. con una norma di portata più generale, si è eliminata per tutte le ipotesi previste dal comma stesso la limitazione dell'esclusione dal patteggiamento ai soli casi di pena superiore a due anni. L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame in Commissione giustizia in seguito all'approvazione di un emendamento presentato dai senatori dell'opposizione, modifica l'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di rito penale, prevedendo che nella formazione dei ruoli di udienza sia assicurata priorità alla trattazione dei procedimenti che vedono coinvolti soggetti che hanno usufruito dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Con l'articolo 8 è stato modificato l'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione di attività di riciclaggio, imponendo l'obbligo di segnalazione anche laddove si sospetti che siano in corso attività di usura. La seconda parte di questo disegno di legge, invece, per la prima volta, introduce nel nostro ordinamento il riferimento alla fattispecie del sovraindebitamento del singolo, dei nuclei familiari e delle imprese non assoggettabili alle procedure concorsuali per passività. Come è noto, la percentuale d'indebitamento delle famiglie italiane in rapporto al prodotto interno lordo è in aumento. La necessità di disciplinare i casi, purtroppo sempre più numerosi anche in conseguenza della grave crisi economica in atto, nei quali il *ménage* familiare risulti economicamente compromesso dallo squilibrio esistente fra reddito disponibile ed ammontare complessivo delle spese ordinarie trova quindi un'adeguata risposta in questo testo legislativo. La nozione di sovraindebitamento, proposta dall'articolo 9, è comprensiva della diversificata realtà di situazioni ad esso in astratto riconducibili. Per sovraindebitamento il disegno di legge intende una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte. Si tratta, in sostanza, di una crisi di liquidità che sorge allorché un *ménage* non dispone, per un certo periodo di tempo, delle liquidità necessarie per far fronte agli impegni precedentemente assunti. Questa crisi di liquidità può essere determinata sia da una variazione negativa dei redditi sia da una variazione positiva delle spese per il consumo. In quest'ultimo caso, la crisi può essere generata anche da spese non ordinarie impreviste che vengono a gravare su di un reddito invariato o addirittura diminuito. Si distingue così un sovraindebitamento attivo, generato dalla crescita delle spese o dalla mancata o inesatta previsione del loro carico sul *ménage* familiare, da un sovraindebitamento passivo, determinato da una crisi reddituale. L'effetto è tuttavia il medesimo: per un periodo di tempo più o meno lungo non si è in grado di assolvere alle ordinarie spese per il consumo, con relativa determinazione di una situazione di crisi che può, per grandi linee, essere accostata a quella che determina il fallimento dell'imprenditore commerciale. Nel caso di debiti cosiddetti non professionali, così dell'individuo come della famiglia, sino ad oggi l'unico strumento disponibile per il creditore era quello dell'ordinario processo esecutivo per espropriazione, il quale nella sua forma tipica presuppone - come è noto - il possesso del titolo esecutivo, quantomeno per il creditore che materialmente assume l'iniziativa del processo. E sappiamo che oggi, per il modo concreto in cui le procedure espropriative, mobiliari e immobiliari, sono regolate nel codice e organizzate nella pratica, ben difficilmente esse giungono ad assolvere una reale funzione di tutela dell'interesse dei creditori. Con il disegno di legge al nostro esame si introduce uno strumento specifico, modellato sulla falsariga di quello fallimentare-concorsuale, per far fronte alle situazioni di crisi sopra indicate, prescindendosi da iniziative del creditore o del ceto creditorio. Molti Paesi europei si sono già mossi in questa direzione: la Francia, per esempio, nel 1989 si è dotata di uno strumento amministrativo e giudiziario volto a regolare il fenomeno del sovraindebitamento (con legge del 31 dicembre 1989); l'Inghilterra dal 1986 ha introdotto una procedura di fallimento civile, diretta da un giudice a ciò delegato, nella quale possono confluire debiti di diversa natura, salvo quelli fiscali ed alimentari; la Repubblica federale tedesca e i Paesi Bassi prevedono strumenti analoghi. Molti altri Paesi, poi, di *common law* (gli Stati Uniti e il Canada, ad esempio) hanno da tempo procedure nell'ambito delle quali, a seconda delle passività accertate, viene favorita la funzione conciliativa tra le parti o la determinazione in via giudiziaria delle condizioni del fallimento civile, sempre con salvezza dei debiti fiscali o alimentari. Gli articoli da 10 a 17 del disegno di legge disciplinano la procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. Un ruolo centrale in questo procedimento svolgono gli organismi di composizione della crisi. Mazzatorta praticamente ad urlare, cosa che non è proprio consona ad un intervento del relatore. *(Brusìo).* Insisto a dire che il relatore dovrebbe poter svolgere la sua relazione in un modo che

il Segretariato sociale, costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera *a*), della legge n. 328 del 2000, gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai. La norma prevede, inoltre, la facoltà per gli enti pubblici di costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità, deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. Per questi soggetti è prevista l'iscrizione in un apposito registro che sarà tenuto presso il Ministero della giustizia. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività loro spettanti, individuati dall'articolo 20, gli organismi di composizione della crisi, che assumono un ruolo centrale in questa procedura, possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 2003. Il testo prevede infine una disciplina transitoria per la quale il Ministro della giustizia dovrà stabilire con uno o più decreti, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente disegno di legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi potranno essere svolti in via esclusiva dai medesimi. Anteriormente a tale data, le stesse funzioni possono essere svolte da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto n. 267 del 1942, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. La Commissione è consapevole del fatto che alcune questioni restano ancora aperte, prima fra le quali quella dell'estensione dell'ammissibilità alle erogazioni del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura anche ai soggetti che non rivestono la qualità d'imprenditore, estensione sulla cui fattibilità è necessaria però un'accurata verifica. Tuttavia, non vi è dubbio che il testo proposto rappresenti uno strumento di notevole efficacia per contrastare gli effetti criminogeni di fenomeni di sovraindebitamento che, con l'acuirsi della crisi economica, appaiono purtroppo sempre più gravi e diffusi. Tenuto conto della sostanziale condivisione registratasi nel corso della trattazione in Commissione, auspico che l'esame in Aula possa essere quanto mai costruttivo e condurre all'approvazione del testo in tempi brevi.

Signora Presidente, spero di utilizzare anche meno dei venti minuti

La Presidenza preferirebbe non essere obbligata ad interrompere la seduta. Prego,

da una cultura dominante fondata sul debito e sul ricorso al credito facile per affrontare un problema o superare difficoltà contingenti, produce un aumento esponenziale del ricorso all'usura.

demarcato nei primi anni '90 dalla privatizzazione del Credito Italiano con lo slogan «Oltre i BOT i Credit», senza spiegare che i titoli di Stato erano a reddito fisso, mentre le azioni presentavano dei rischi. Siamo passati ad essere un popolo di debitori, specie nel passaggio dalla lira all'euro nel 2002, che ha provocato un raddoppio dei prezzi ed un'enorme speculazione a danno delle famiglie, sempre più a rischio di indebitamento. Stime recenti riferiscono di un rischio di sovraindebitamento proiettato nel 2009 che, soprattutto nel Mezzogiorno, toccherebbe 464.000 famiglie e 570.000 piccoli imprenditori. Il debito medio delle famiglie nel Sud raggiungerebbe i 22.000 euro, quello dei piccoli imprenditori i 40.000 euro; cifre che, se confermate e valutate alla luce della scarsa propensione delle banche ad elargire credito, richiedono un deciso intervento pubblico sul fronte del microcredito "sociale", anche in chiave di prevenzione rispetto al fenomeno dell'usura, rispetto alla cui diffusione il numero di denunce presentate all'autorità giudiziaria non dà una misura attendibile della reale entità dei problemi. Nell'ordinamento giuridico l'usura è stata annoverata tra i delitti solo dal 1931, con l'introduzione del codice Rocco, nel quale si pose un limite all'interesse che il creditore poteva vantare nei confronti del debitore; una nuova normativa, la legge ha inasprito le pene a tutela delle vittime dell'usura. Oggi l'Occidente è in balia di poche famiglie che comandano l'industria petrolifera, le banche e, tra le attività illecite più remunerative, il traffico d'armi e il commercio della droga. Della tradizione biblica e delle sue norme morali, che impedivano ad un capitale la produzione di interesse, non resta più nulla. La legge n. 108 del 1996 vide la luce dopo l'impegno e la mobilitazione di cittadini e piccoli imprenditori strozzati dalle banche. Bisogna sapere che gran parte dell'usura nasce in banca, da un credito rifiutato, da un rientro inspiegabile di un fido. Quindi, nel 1996, con l'appoggio di uomini di Chiesa, da monsignor Di Liegro a padre Rastrelli, alcune associazioni fecero presentare un testo mutuato dalla legge francese a Camera e Senato. Ci ricordiamo il «Treno contro l'usura» della Confesercenti per arginare lo strapotere di istituti di credito che, oltre ai tassi applicati su prestiti ed impieghi bancari, praticavano l'anatocismo (ovvero la capitalizzazione trimestrale degli interessi), con una maggiorazione della commissione di massimo scoperto, quel vero e proprio pizzo legalizzato che ho denunciato più volte in quest'Aula. Questo disegno di legge, che il Senato si accinge a votare dopo un approfondito esame condotto dalla Commissione giustizia con spirito costruttivo e di collaborazione tra i diversi schieramenti politici, consente di affrontare con la dovuta rilevanza un tema di grande attualità. L'usura è da sempre, ma ancor di più lo diviene in tempi di crisi economica e finanziaria quali gli attuali, una piaga sociale che trova terreno fertile nello stato di povertà e di indebitamento delle famiglie. Viene quindi in rilievo, al di là degli interventi lodevoli che stanno alla base del disegno di legge e della sua formulazione, una realtà sottostante che suscita allarme sociale, in particolare nelle realtà del Mezzogiorno più fortemente colpite dalla crisi. mesi del 2009, è cresciuto di quasi il 70 per cento. Il passo dal sovraindebitamento all'usura non è automatico o inevitabile, in quanto i dati rilevano come la maggioranza delle famiglie sovraindebitate non evolva nell'usura; è altresì vero che in moltissimi casi di usura si riscontra una lunga fase di indebitamento precedente al fenomeno usurario. Se il nesso lineare tra sovraindebitamento e usura non consente di valutarne una relazione in stretti termini di consequenzialità, resta assodato che si tratta di un percorso complesso, implicante una serie di fasi storico-temporali durante le quali i diversi attori coinvolti (la famiglia, la rete sociale, le istituzioni, gli istituti di credito) conoscono una fase di sovraindebitamento che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni assunte. Negli ultimi cinque anni i debiti delle famiglie risultano aumentati in media del 40 per cento, con punte massime che superano il 50 per cento in alcune province. E se anche i dati raccolti all'inizio del 2009 non confermassero la crescita del debito, ci si troverebbe di fronte ad una conseguenza della contrazione dei consumi,

nell'entroterra di Genova, un geometra che aveva perso il lavoro è stato ritrovato impiccato; qualche giorno prima, altri che avevano perso la casa, perché non potevano pagare le rate del mutuo, hanno fatto la stessa fine. Uno dei meriti del disegno di legge in esame consiste nel portare alla luce un fenomeno, quello del sovraindebitamento, pressoché ignorato dai tanti decreti‑legge anticrisi. Al contempo, uno dei limiti di questo disegno di legge è quello di affrontare il problema dal punto di vista eminentemente "tecnico" e in un'ottica strettamente procedimentale, come peraltro era inevitabile. l'azione del Governo resta, a nostro avviso, fortemente carente, tutta orientata come è all'erogazione di fondi per la grande impresa o i grandi istituti di credito, mancando di visione strutturale e di intervento sistematico sui redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e sul sostegno al reddito di quanti non hanno lavoro o, avendolo, lo perdono senza disporre di una rete di ammortizzatori sociali. Lo stesso disegno di legge in esame, che nel testo inizialmente presentato dal senatore Centaro faceva riferimento espresso e privilegiato alle famiglie come centro di riferimento, si è venuto trasformando in un Capo II che, ampliando la nozione di "debitore" cui riferire le nuove procedure di concordato, rischia di far scomparire al suo interno la realtà vissuta da migliaia di famiglie in difficoltà economica. Questi nuclei, siano essi famiglie numerose come monoparentali, vivono una realtà di crisi, non tanto per la contrazione congiunturale del giro d'affari aziendale, quanto piuttosto rispetto ad una realtà quotidiana che li vede in rapporto con il proprietario di casa per il canone di affitto, piuttosto che con la finanziaria per il rateo connesso all'acquisto di un'automobile, ovvero con la banca per i mutui connessi all'acquisto o alla ristrutturazione della propria casa. Non stiamo quindi parlando di spese voluttuarie, bensì di una crisi di debito che investe spese necessarie e basilari. Nel Capo I del disegno di legge in esame sono previste alcune modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione che potrebbero essere integrate con un rafforzamento della parte pecuniaria delle sanzioni, alla luce del carattere ormai "industriale" ed organizzato che molti fenomeni di usura presentano. In tal senso, è stato positivo l'intervento della Commissione sull'articolo 629 del codice penale, mentre un innalzamento della sanzione pecuniaria, soprattutto nel massimo, per lasciare un giusto ambito di apprezzamento al giudice potrebbe essere utile, anche con riferimento all'articolo 644 per l'usura propriamente detta. Con il Capo II viene introdotto un nuovo procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, che rappresentano una delle ragioni del ricorso al mercato dell'usura. Appare opportuno in questo Capo introdurre alcune cautele rispetto ai requisiti oggettivi dei beneficiari, parallele e ulteriori rispetto a quelle che la Commissione ha voluto porre nel Capo I circa la concessione dei prestiti. Con riferimento all'usura nella quale il sovraindebitato può incappare, troviamo un quadro "ufficiale" piuttosto rasserenante e uno scenario "reale" più confuso e inquietante, sui quali le istituzioni rischiano di contraddirsi, visto che in molte realtà territoriali lo strumento dell'Osservatorio antiusura e antiracket è rimasto sulla carta. Di qui, la situazione paradossale che si registra in alcune aree del Paese. Si conviene con l'articolo 2, che precisa il concetto di evento lesivo, presupposto essenziale per l'elargizione a favore dei soggetti vittime di attività estorsive, consentendo la cumulabilità con provvidenze provenienti da altre amministrazioni e con gli articoli 4 e 5, che prevedono rispettivamente l'aggravante di pena, anche nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari e l'affidamento al giudice della decisione di restituire o meno i titoli, i beni e le utilità sequestrati all'indagato, in caso di estinzione del reato di usura. Mi accingo alla conclusione, signora Presidente, e per non annoiare, se me lo consente, depositerò

giustizia si dice consapevole del fatto che resta aperta la questione di un'estensione dell'ammissibilità dell'erogazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estortive e dell'usura anche ai soggetti che non rivestono la qualità di imprenditore.

che quelle famiglie che avevano un debito del genere possano essere iscritte in queste banche dati che sono di origine privata e non della Banca d'Italia, come dovrebbe essere, perché a seguito di tutti i rubinetti del credito. Mi auguro quindi che l'emendamento 21.202, che intende porre dei tetti alle segnalazioni presso le centrali rischi private, in uno spirito *bipartisan,* perché tutti, maggioranza ed opposizione, dovremmo avere a cuore le sorti delle famiglie, di quei lavoratori che si debbono impiccare perché perdono il posto di lavoro, di quelle persone cui

Signora Presidente, onorevoli colleghi, la normativa vigente in materia di lotta all'usura e all'estorsione, pur avendo il merito di aver dato una risposta concreta ai problemi legati a tali fenomeni criminali, evidenzia oggi punti di debolezza, tanto da far emergere la necessità un nuovo intervento legislativo. L'usura rappresenta un problema socialmente rilevante e meritevole di un'attenzione costante e vigile. Proprio per questo ho ritenuto necessario presentare in data 25 settembre 2008 il disegno di legge n. 1056, indicante norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione. Ringrazio pertanto il presidente della Commissione giustizia Berselli, il relatore

307 del collega Centaro, che trattava la materia in una visione certamente più ampia e approfondita. In Italia il problema dell'usura è stato affrontato prevalentemente cercando di attivare metodologie di prevenzione, peraltro concentrate quasi esclusivamente nelle zone del Sud d'Italia, come dimostrato dagli interventi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999 n. 44. Tuttavia l'usura non è un fenomeno circoscritto a tali aree; al contrario, è presente in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, pur caratterizzandosi con peculiarità diverse, ed investe soprattutto le aree produttive ad alto sviluppo del nostro Paese. Nella lotta all'usura va detto che le associazioni e le istituzioni antiusura e antiestorsione riconosciute, di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996, hanno avuto un ruolo determinante. Tali associazioni, da più di dieci anni, sono impegnate con successo nelle attività di prevenzione e lotta all'usura e all'estorsione, nonché in attività di assistenza e solidarietà nei confronti dei soggetti danneggiati dalle attività estorsive; ciò a dimostrazione del fatto che nella lotta a tali fattispecie di reato il fattore associativo risulta vincente. In tale contesto, appare opportuno favorire lo sviluppo dell'associazionismo al fine di meglio combattere i fenomeni di criminalità organizzata, distinguendo le diverse capacità e rappresentatività territoriali. La modifica dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, prevista dal mio disegno di legge e inserita nel nuovo testo, valorizza l'esperienza e le professionalità maturate negli anni da tali associazioni, recependo in pieno il principio di sussidiarietà, favorendo così l'azione del *non profit*; principio di sussidiarietà che vorremmo sempre alla base delle nostre azioni politiche. Come ricordato dal relatore e anche dal collega Lannutti nel suo intervento, molto preciso e puntuale, una questione che resta ancora aperta è quella appunto di ampliare l'accesso al Fondo di solidarietà anche a soggetti che non rivestano la qualifica di imprenditore. Infatti la citata legge n. 108, all'articolo 14, non prevede ancora interventi a favore di percettori di reddito, dipendenti, famiglie e pensionati, ma solo a favore di soggetti produttori di reddito. Ci auguriamo appunto che il dibattito e l'azione del Governo nel tempo possano colmare questa lacuna trovando le risorse necessarie. Diparticolare importanza ritengo, inoltre, il Capo II del disegno di legge che introduce un nuovo e importante istituto, il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, il quale è volto a porre rimedio alle situazioni di sovraesposizioni economiche che rappresentano una delle ragioni più frequenti del ricorso al mercato dell'usura. Ritengo che proprio questo Capo II, l'intuizione di intervenire con questo nuovo istituto e l'articolazione prevista, sia uno dei punti salienti e caratterizzanti il testo legislativo in esame e che possa veramente andare verso un'azione di composizione di tutte quelle piccole e medie vertenze che forse con tale istituto potranno trovare una sintesi e una risoluzione importante. Concludo, onorevoli colleghi, con un doveroso e meritato plauso per questa iniziativa legislativa e per l'approfondito lavoro svolto in Commissione, che interviene con efficacia e tempestività su un fenomeno come quello dell'usura che nel momento di crisi economica attuale, se non contrastato con forza e determinazione, potrebbe dilagare nei suoi effetti criminogeni, trovando terreno fertile nel rischio di sovraindebitamento delle famiglie italiane.

questa è una situazione paradossale ed insostenibile. Noi chiediamo quindi con forza - questo è un punto per noi molto importante - che di questo venga data comunicazione al soggetto, in modo che possa innanzitutto rendersene conto

noi possono migliorare ulteriormente il testo all'esame dell'Aula.

sia nella situazione economica attuale, cioè nella crisi, sia rispetto al fenomeno della criminalità organizzata. La recessione economica costituisce in questo momento un'opportunità per la criminalità organizzata, soprattutto per la mafia, di arricchirsi, favorendo aumento di estorsione e, soprattutto, soprattutto, di usura. Di fronte alla chiusura dei canali di credito da parte delle banche, commercianti e imprenditori troveranno chiaramente come principale finanziatore le mafie, che hanno la necessità di riciclare grandi quantità di denaro. È un discorso inevitabile, perché la diminuzione del credito legale fa aumentare quello illegale, garantito da usurai e mafiosi. La mafia, a differenza dell'usuraio semplice, non è interessata a portare alla disperazione l'usurato, quanto piuttosto alla sua azienda, che le serve per investire e ripulire il denaro. E l'imprenditore in crisi, dopo aver ceduto l'azienda alla mafia, così salvandola dalla bancarotta, può diventare un dipendente a sua volta dell'organizzazione mafiosa, tanto che potrà addirittura guadagnare più di prima, perché rilevato dall'organizzazione ed emancipato perfino dal rischio d'impresa. È chiaro che il comune interesse economico fa, insieme, dilagare e rendere molto da scoprire il fenomeno del riciclaggio. L'usura tuttavia è in agguato anche per milioni di famiglie italiane che rischiano di esserne vittima al pari delle piccole imprese, che già hanno subito gli effetti della crisi economica. Secondo le associazioni antiusura, il debito a lunga scadenza, per essere chiari il mutuo, che attiene soprattutto alle abitazioni, costituisce il problema più urgente, al pari degli atteggiamenti persuasivi delle società di recupero credito. I dati riportati dalla stampa ci danno una diffusione dello stato di povertà delle famiglie italiane che colpisce soprattutto le Regioni meridionali, proprio quelle a maggiore presenza di organizzazioni mafiose, sempre pronte a reclutare manovalanza in danno dello Stato. L'allarme viene dato dalle associazioni dei consumatori, che lamentano il sovraindebitamento delle famiglie del Mezzogiorno nei primi due mesi del 2009. I dati forniti dall'Associazione contribuenti italiani, che monitora il fenomeno in Italia, parlano di un sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole imprese con una crescita del 69,4 Il rischio per le famiglie del Mezzogiorno è preoccupante secondo le denunce delle associazioni. Si parla di 464.000 famiglie e di 570.000 piccoli imprenditori a rischio. Al primo posto la Sicilia. Seguono Campania, Puglia, Calabria e, per ultime, Basilicata e Molise. Il rischio reale è quindi che molte famiglie ed imprese del Meridione possono cadere nelle mani di usurai più o meno collegati alla mafia. Ma il problema viene denunciato anche in altre aree d'Italia, tanto che in Piemonte l'Associazione contribuenti italiani lancia un allarme per 394.000 famiglie piemontesi a rischio di povertà, con una situazione concorrenziale rispetto perfino alla Sicilia e alla Campania. Quindi le richieste di aiuto agli sportelli Confesercenti crescono del 20‑30

recente il ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni, in una conferenza stampa ha dichiarato che nel clima di crisi economica nel Lazio si registrano più casi di usura, ma contemporaneamente un basso numero di denunce e di accesso delle vittime al Fondo di prevenzione, aggiungendo che, nel corso della riunione tenutasi con la giunta dell'Unione degli industriali e delle imprese di Roma, era stato segnalato che "nel Lazio e a Roma si concentrano tutte le organizzazioni criminali strutturate in Italia". Per questo, oltre ad agire sul Fondo di prevenzione dell'usura gestito dal Ministero dell'economia, egli aveva chiesto agli imprenditori di collaborare e denunciare "fenomeni che presumibilmente si aggravano in momenti di crisi economica".

tracciamento e, ove possibile, di videosorveglianza. Inoltre, per colpire le basi economiche della mafia e sradicare il processo di conquista

appartenenti anche al settore del credito, attraverso cui si radica la potenza della mafia e quindi implementare la lotta a tutti quei reati strumentali che non sempre possono essere inquadrati nella criminalità mafiosa in senso stretto: ciò vale dunque anche per l'usura e l'estorsione. In particolare, per quanto riguarda le estorsioni, fattispecie che in qualche maniera è toccata dal provvedimento che ci accingiamo ad approvare, vorrei ricordare che la mafia gestisce tale attività soprattutto nei territori in cui ha un controllo primario, in cui esercita cioè un controllo del territorio e in cui l'imprenditore è sempre a conoscenza della qualità del soggetto che gli fa la richiesta. Tuttavia, la mafia può avere interessi e capitali in anche se non è fisicamente presente. Per tale motivo i soldi della mafia prima o poi richiedono la presenza e i metodi dei mafiosi; di conseguenza, l'estorsione, come l'usura, si estende a estende a tutte le altre Regioni d'Italia e colui che paga, accettando forme di controllo, finanzia la mafia e quindi la fa crescere. Di fronte a questa situazione nessuno può sottrarsi: il Parlamento, il Governo le pubbliche amministrazioni, gli istituti di credito, le imprese e i privati cittadini. Per combattere la crisi occorrono risposte adeguate: innanzitutto da parte del Governo, che parallelamente dovrà non solo rafforzare e curare l'economia e la sofferenza che in questo momento investe gli italiani, ma soprattutto pretendere e imporre il rispetto della legalità e la solidarietà di una comunità completa, ovvero di tutto lo Stato italiano. Stato italiano. Nel disegno di legge in esame alcune risposte vengono offerte: nella relazione, il senatore Mazzatorta ha messo in luce come la Commissione sia consapevole del fatto che alcune questioni tecnico-giuridiche restino aperte: tra queste è sicuramente aperta quella della platea dei possibili destinatari dei benefici, a cui hanno accennato alcuni colleghi in precedenza. Condivido pienamente questa impostazione, ma ritengo sia giusto aggiungere che restano da affrontare con la massima

tra l'altro, serve a ridurre gli oneri finanziari connessi al programma di protezione in pendenza del procedimento penale ovvero gli stessi oneri derivanti dalla concessione dei benefici del Fondo di solidarietà.

usurari; non solo per il maggior disvalore penale della condotta, ma anche per potere anticipare la soglia di rilevanza penale rispetto a tale tipo di comportamenti. La tutela delle vittime dell'usura è stata rafforzata con la possibilità di ottenere l'erogazione dei mutui da parte del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura anche da parte dell'imprenditore individuale dichiarato fallito che non sia stato condannato per bancarotta semplice o fraudolenta o per altri delitti di indole patrimoniale. Parallelamente, si è deciso quindi di escludere dalla possibilità di ottenere erogazione di mutui soggetti che siano stati condannati per delitti di usura, criminalità organizzata o reati per i quali l'arresto fragranza sia obbligatorio, nonché coloro cui siano state applicate misure di prevenzione personali o patrimoniali. Al di là dell'estensione della categoria dei beneficiari delle elargizioni per soggetti danneggiati da attività estorsive, che ancora richiede qualche aggiustamento, è particolarmente importante la previsione di appositi procedimenti, come già ricordato da alcuni colleghi, per la composizione della crisi da sovraindebitamento: è sicuramente l'aspetto più rilevante del provvedimento, in quanto si prevede che ogni qual volta il debitore sia impossibilitato ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, possa proporre ai creditori un accordo. Inoltre, è possibile integrare il patrimonio del debitore e la proposta di concordato verrà sottoposta ad una rigida valutazione da parte del giudice, nel corso della quale potranno intervenire i soggetti interessati. Anche al prefetto vengono attribuiti compiti particolarmente importanti. Al fine di evitare frodi da parte del sovraindebitato, si è voluto attribuire rilevanza penale ad alcune condotte di dolosa alterazione della massa patrimoniale da parte del debitore.

Quindi, va collegata al racket estorsivo, al riciclaggio e a quelle contraddizioni del nostro sistema economico-finanziario che alimentano direttamente e indirettamente la dilagante patologia dell'usura. Il disegno di legge costituisce un passo avanti proprio in tale direzione quanto affronta per la prima volta la questione dell'usura in una chiave di sistema. Mi riferisco direttamente al problema del sovraindebitamento e le esperienze legislative degli altri Paesi europei hanno dimostrato la difficoltà nell'applicazione delle misure del concordato. Sarà la realtà ad incaricarsi di verificare come questa procedura possa essere agilmente applicata. L'altra positività di questo disegno di legge, ed è merito del senatore Centaro, è di aver proposto norme che recepiscono la prassi consolidata del Comitato per la solidarietà alle vittime del racket e dell'usura. Faccio un solo esempio, quello relativo all'imprenditore fallito che nella prassi del Comitato era stato già risolto e superato. e superato. Al di là di questa positività, lo stesso relatore, senatore Mazzatorta, confessa che l'intervento è parziale. è parziale. E lo è perché per poter essere un intervento definitivo non deve soltanto essere collegato alla questione criminale, ma anche alle contraddizioni del nostro sistema economico‑finanziario. Ne cito solo alcune. Innanzitutto, come è possibile che ancora oggi (se non per la difesa di apparati ministeriali) ci sia da un lato un Fondo di solidarietà e dall'altro un Fondo per la prevenzione,

fondazioni e dei confidi sia un'attività di minor valore, mentre la visione del sistema pubblico di prevenzione e di solidarietà dovrebbe essere unitario. Abbiamo pertanto un apparato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro presso il Ministero dell'interno sotto la responsabilità del Comitato presieduto dal Commissario straordinario. È inutile effettuare prelievi, basterebbe una sola autorità destinataria di entrambe le funzioni, di prevenzione e di solidarietà, per rendere più incisiva e reale la risposta ai cittadini che hanno avuto il coraggio di denunciare l'estorsione e l'usura e che hanno necessità di ricevere risposte immediate dallo Stato per uscire dal tunnel della loro disperazione che spesso porta al suicidio. E vengo alla seconda contraddizione del sistema.

il tasso soglia, un tasso mai secondato, quando non rispettato, da misure adeguate per colpire l'usura bancaria. E come è possibile che sia previsto un tasso soglia per il sistema bancario, mentre le finanziarie - spesso espressione dei gruppi finanziari - arrivano a praticare, con dei sistemi e delle tecniche di rinnovo trimestrale, fino al 60 per cento di interesse su base annua?

che prevedeva, per le vittime del racket e dell'usura che avessero denunciato, la non interruzione dei fidi, cosa che invece si verificava puntualmente ogni qual volta una notizia di stampa locale metteva in evidenza che una vittima aveva denunciato. Immediatamente la banca ritirava.

anche di 100 euro, venivano gettati nelle mani della rete criminale degli usurai. Questo, quando non ci sono bancari infedeli, specie nel Mezzogiorno d'Italia, che sono direttamente collegati alle reti degli usurai e della criminalità e muovono il fido a loro piacimento, anche in rapporto ai flussi di cassa delle piccole e medie aziende, e spingono direttamente

che compie una radiografia accurata dei sistemi di occultamento del riciclaggio e del rapporto tra usura, estorsione e riciclaggio.

specializzate nelle fideiussioni, sono le principali riciclatrici di denaro sporco. Quando si affronta, allora, il problema della pubblicità ingannevole?

e che ancora una volta richiamano il Parlamento ad un'attenta capacità di intervenire in modo mirato, facendo tesoro dell'esperienza maturata in questi anni e, nello stesso tempo, cercando di risolvere alcuni nodi irrisolti che ci trasciniamo e che non abbiamo mai avuto il coraggio di affrontare direttamente.

Ecco perché abbiamo assunto un atteggiamento positivo su questo disegno di legge. I nostri colleghi hanno offerto un contributo prezioso all'interno della Commissione giustizia. Da parte del Partito Democratico c'è stata una piena e sincera collaborazione; il relatore ha dato atto che alcuni emendamenti hanno arricchito il disegno di legge, ma naturalmente manteniamo una nostra autonomia di analisi e siamo pronti ad avanzare altre proposte, che in questo disegno di legge non affrontiamo, per fare quel grande salto di qualità che oggi ci viene richiesto nella lotta alle estorsioni, ai vari sistemi di usura. Colleghi, sapete bene che le mafie non possono fare a meno delle estorsioni: con le estorsioni si assicurano un fitto e garantito controllo del territorio; grazie alle estorsioni sono in grado di sapere e di capire cosa avviene in quella via, in quel quartiere, in quella città, in quella comunità e sanno anche immediatamente coglierne l'evoluzione: chi apre e chi chiude, chi cresce, chi va indietro. sono in grado anche di accumulare ingenti risorse per il pagamento delle spese legali, che in questa fase storica, grazie all'azione dello Stato, grazie alla positiva irruzione del giudizio penale all'interno del nostro sistema democratico, con processi, indagini e condanne, sono sempre più ingenti nel nostro Paese. Con le estorsioni riesce a sostenere il pagamento delle spese legali, preziosissimo per le organizzazioni mafiose. garantiscono un reddito all'interno delle casse delle organizzazioni mafiose per alimentare una sorta di *welfare* per mantenere le famiglie dei mafiosi. Quando una famiglia mafiosa subisce l'arresto del proprio capo ecco che immediatamente subentra il sostegno al reddito dei suoi esponenti, e così, attraverso quell'entrata, c'è un'immediata risposta ad una possibile crisi che si potrebbe aprire; allora si tappano le bocche, si crea omertà, si crea quella fitta rete di integrazione in grado anche di assorbire e superare possibili crisi, come possibili potenziali forme di collaborazione con la giustizia.

le proprie abilità, la propria capacità di saper individuare quale deve essere il rapporto qualità‑prezzo verso il quale orientare le forniture come gestire la competizione, la concorrenza, come poter migliorare il proprio apparato produttivo. Infine, attraverso le estorsioni, si alimenta il sistema delle collusioni con settori dell'economia, perché attraverso di esse, soprattutto negli appalti pubblici, le organizzazioni mafiose sono in grado di rovesciare il meccanismo che si crea quando,

pronta ad avere un vantaggio, pronta a mettere a disposizione, oggi, una cosiddetta offerta d'appoggio e, domani, ad essere direttamente favorita nell'aggiudicazione dell'appalto, e magari ancora, quando si hanno difficoltà ad accedere direttamente alla gara, a gestire concretamente con i subappalti in quel cantiere l'attività di quell'opera pubblica. Ecco perché noi dobbiamo fare i conti con il sistema delle estorsioni; non considerarla una funzione marginale della forza, del potere e del controllo delle organizzazioni mafiose, ma farne una sfida, sfida, una scelta qualificata. Così anche sull'usura, cari colleghi. Una pratica odiosa, silente, sommersa, ma forte e devastante; appannaggio, certo, di una larga fascia di criminalità diffusa.

funzione aggiuntiva delle diverse forme di accumulazione mafiosa. Colleghi, con la legge n. 108 del 1996 e la legge n. 44 del 1999 il Parlamento diede una prima e qualificata risposta. per il Parlamento il lavoro, l'esperienza e la fatica delle associazioni antiracket, guidate da Tano Grasso. Grazie a quel lavoro si riuscì in Parlamento a produrre una prima legislazione in grado finalmente di affrontare alcuni nodi;

Quando si è minacciati, lo Stato interviene. Quando si è danneggiati, lo Stato interviene. Quando si è impediti nella propria attività imprenditoriale, lo Stato è in grado di far riprendere il cammino. Si riuscì anche a spezzare il meccanismo della solitudine, facendo in modo che con la denuncia, attraverso il veicolo delle associazioni e attraverso la promozione dell'associazionismo antiracket, si potesse finalmente lasciare

potenza. Sul versante antiusura sono state preziose anche le esperienze e le microrealtà che si sono autorganizzate, dall'educazione all'uso corretto del denaro fino a garantire, attraverso le prime forme di consorzio, quel bisogno di credito che spesso il sistema bancario negava, umiliava e addirittura, in molti casi, orientava verso gli usurai. Cari colleghi, si è trattato di una legislazione sicuramente positiva; essa, attraverso l'esperienza dei vari commissari nazionali antiracket o antiusura, si è potuta consolidare e diffondere su tutto il nostro territorio. Ma oggi abbiamo alcuni nodi irrisolti. Penso, ad esempio, alle squadre investigative specializzate, alla necessità di garantire percorsi particolari nell'organizzazione dei processi, per fare in modo che i processi di racket e di usura trovino quella risposta veloce che spesso ci viene indicata

dell'accesso al credito un punto di forza di un Paese avanzato, in grado di valorizzare la capacità imprenditoriale delle piccole e medie imprese, e non, viceversa, un sistema vincolistico. In questo particolare momento di crisi, nonostante tutti gli annunci che vengono fatti, nonostante l'utilizzo dei cosiddetti Tremonti *bond*, sappiamo che nella pratica quotidiana c'è una richiesta di rientro spietata, che non tiene assolutamente conto della qualità del progetto e dell'iniziativa imprenditoriale, o di una particolare difficoltà imprenditoriale, ma tiene conto soltanto di quella antica, barbara e classica capacità patrimoniale delle singole persone che sono impegnate a vario titolo nell'esercizio dell'attività di impresa. Ecco perché con questi nodi irrisolti dobbiamo fare i conti: in questa fase di crisi, in cui l'espansione dell'attività delle mafie rischia paradossalmente di crescere, anche in costanza dei grandi successi che abbiamo ottenuto in questi mesi

al tema della denuncia obbligatoria, al quale giriamo intorno, senza affrontarlo, perché non tentiamo di trovare la soluzione più adeguata, ma piuttosto pensiamo di saltare complessivamente questo ostacolo, che potrebbe trasformarsi in una grande risorsa di libertà, di competizione e anche di resistenza da parte delle imprese. potrebbe innescare l'idea di una denuncia obbligatoria di fronte ad imprese che oggi sono pronte, che sono magari più disponibili di una volta, come hanno dimostrato gli imprenditori della Confindustria siciliana e delle tante associazioni antiracket nate anche in questi mesi.

la singola soggettività dell'imprenditore mafioso, ma un altrettanto oggettivo interesse dell'imprenditore a non pagare e a dimostrare all'organizzazione mafiosa che questo non è solo il frutto della sua parziale

delle varie organizzazioni mafiose. Se questo lo applicassimo almeno nel sistema degli appalti, pensate che benefici avremmo nel liberare il mercato dal vincolo delle organizzazioni mafiose, nello stabilire dove si devono pagare

nel poter resistere, al di là del controllo esterno che le forze dell'ordine possono fare su quanto avviene concretamente e quotidianamente, che alla fine invece sposta sempre più la forza dell'imprenditore verso l'assoggettamento all'organizzazione mafiosa.

invece la forza di recupero nella lotta al riciclaggio è molto bassa, piccolina, con percentuali che non superano neanche l'1 o il 2 per

pochissimi risultati e molto parziali. Piuttosto che aspettare a valle che l'operazione sospetta si compia per poi affidarci alla responsabilità degli operatori, dobbiamo andare a monte e fare della tracciabilità del denaro la forza di un'economia aperta, libera e trasparente. La tracciabilità del denaro è infatti la frontiera più avanzata su cui si può organizzare una moderna lotta alla mafia che possa coniugare legalità e sviluppo, libertà d'impresa e rispetto delle regole di mercato.

in processi e in indagini di mafia possano usufruire di queste provvidenze importanti, che devono diventare una risorsa per premiare chi denuncia, chi resiste e si sottrae al sistema di ricatto e di collusione mafiosa.

e su altri tipi di intervento. Infine, sottolineo la positiva capacità di individuare un insieme di norme insieme di norme riguardo al sovraindebitamento, un meccanismo che in questa fase di crisi crea dei problemi serissimi al mondo dell'impresa e lo trascina in condizioni disperate verso la chiusura e il fallimento.

l'attività imprenditoriale, farla vivere, darle la possibilità di superare le crisi e fare in modo che il superamento della crisi diventi un successo da parte dello Stato.

ad affrontare, su cui siamo disponibili ad offrire quell'elaborazione che non è solo nostra, ma è pronta nella società ed è in grado finalmente di ottenere i successi che tutti ci aspettiamo nella lotta al racket e all'usura.

il problema perché non ricevono lo stipendio dal mese di dicembre e neanche l'indennità di cassa integrazione.

Si tratta di una figura professionale estremamente importante anche perché, purtroppo, l'assistenza psicologica nel nostro Paese si limita ad uno o due interventi per detenuto e ciò, in parte, a causa del sovraffollamento delle carceri, in parte, a causa della scarsa disponibilità di psicologi. Questo determina purtroppo fenomeni gravi di autolesionismo, che sfociano in alcuni casi anche nel suicidio, com'è accaduto nella mia città tre giorni fa. Il sottosegretario Caliendo mi ha assicurato che l'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della giustizia stanno cercando una soluzione a questo problema, che può essere transitoria come definitiva,

Signora Presidente, per quanto concerne gli psicologi, si tratta di un concorso ultimato nel 2006: fu approvata la graduatoria, ma i vincitori non furono assunti per mancanza di fondi.

Questa è la situazione; noi non abbiamo più possibilità d'intervenire, se non in questa limitata forma.

La seduta è tolta